L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente,

onorevoli senatori, nella seduta di ieri la Commissione affari costituzionali ha esaminato il disegno di legge n. 953,

di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA». Chiederei ai colleghi di prendere posto in modo tale da consentire al presidente Bianco di svolgere la sua esposizione. Prego, Presidente. BIANCO *(Ulivo)*.

Dopo una esposizione del senatore Villone, relatore alla Commissione, che proponeva un parere favorevole, è intervenuto nel dibattito il senatore Pastore, motivando un dissenso più di prospettiva sulla soluzione a regime della vicenda connessa alla sentenza europea che riferito al decreto in sé considerato. Nondimeno, legittimamente l'opposizione si è orientata per un voto di astensione alla proposta di parere favorevole, con l'eccezione del senatore Palma che ha annunciato il suo voto contrario. All'atto della votazione, la proposta di parere favorevole raccoglieva dieci voti positivi, nove astensioni e un voto contrario. Data la parità di voti tra favorevoli e non, la proposta di parere risultava non approvata, cosicché, in ragione della peculiare natura dei pareri della 1a Commissione sui presupposti costituzionali dei decreti-legge, che sono fondati su un criterio rigorosamente binario (i presupposti sussistono o meno), l'esito dell'esame è stato quello di un parere negativo, che oggi viene sottoposto all'Assemblea ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, siamo in una situazione che è abbastanza rilevante perché noi, come Unione, in Commissione non siamo riusciti a garantire la nostra partecipazione di maggioranza. Tuttavia, vorrei rilevare come i presupposti di costituzionalità e di urgenza siano stati ammessi dallo stesso rappresentante della Casa delle Libertà; quindi abbastanza capzioso che ora, di fronte all'attuazione di una sentenza di cui il Governo prende atto con urgenza con un decreto, su una tematica che dovrebbe stare a cuore, almeno a quanto leggemmo allora e leggiamo tutti i giorni, ai rappresentanti della Casa delle Libertà, pur di fare un piccolo passo verso quell'ambiente che veniva richiamato dalla Capogruppo dell'Ulivo stamattina, sia disposti ad ostacolare in tema di costituzionalità e di urgenza un decreto che è doveroso e necessario e che dovrebbe poiché ovviamente ne sono tutt'altro che convinto - andare in direzione del famoso "popolo dell'IVA", dando cioè garanzia ai contribuenti che, con questo decreto, avranno la sicurezza di poter avere il rimborso di quanto versato relativamente all'IVA. potremmo trovarci di fronte, senza il compatto voto dell'Unione, ad un decreto che decade per volontà della Casa delle Libertà, complicando, quindi, un percorso che, dopo la sentenza europea, è un diritto di questi cittadini.

credo che il voto di astensione pronunciato in Commissione dal centro-destra sia pienamente legittimato anche sul punto dell'urgenza,

dell'IVA degli autoveicoli per le imprese ed i professionisti: nessuno ha messo mano a tale importante segmento della normativa IVA nazionale e, prima o poi, doveva arrivare questa che possiamo considerare, in maniera*bipartisan*, una tegola per le nostre finanze pubbliche.

di segnalarlo ai colleghi qui in Aula. In primo luogo - com'è noto - le sentenze della Corte di giustizia non cancellano dal nostro ordinamento le norme illegittime,

gli imprenditori ed i professionisti che hanno vissuto in tale contesto normativo di indeducibilità da domani si troveranno in una situazione, direi, paradossale

non applicandole potrebbero ottenere comunque (attraverso la Corte di giustizia o, ancor prima, i giudici nazionali, che si adeguerebbero alla giurisprudenza di questa) il rimborso delle somme legittimamente pagate. E cosa faranno i nostri operatori? Certamente dedurranno l'IVA in spregio alla norma scritta, ma avranno un contesto formale di effettiva, apparente illegittimità.

di rispettare il dettato formale della legge oppure di non rispettarla affatto, trovandosi magari l'indomani in una situazione di illegalità. Allora, questo decreto-legge non fa quello che avrebbe dovuto fare: rimodulare, rimodellare, riscrivere la normativa IVA e dare certezza per il futuro delle nostre imprese e dei professionisti, cioè di tutto il settore del lavoro autonomo. Ma fa qualcosa sulla quale si può esprimere una valutazione di censura: di censura: si preoccupa solo di limitare, di ridurre, di depotenziare quello che è, in base alla sentenza della Corte di giustizia, l'esercizio sacrosanto di un diritto al rimborso.

termini perentori, ricorso a modulistiche e, soprattutto, con la non applicabilità in questo settore delle norme relative alla detrazione e alla compensazione dell'imposta sul valore aggiunto non detratta a suo tempo e quindi pagata in maniera illegittima. Signor Presidente, riconoscendo le difficoltà trova, si è trovato e si troverà qualsiasi soggetto, qualsiasi forza politica, qualsiasi coalizione che deve riaffrontare e risolvere questo problema, a noi sembra che il decreto-legge in esame sia assolutamente insufficiente per quanto riguarda il futuro del settore normativo dell'IVA

era ed è necessaria, nello stesso momento in cui il decreto viene emesso e mi meraviglio di come questo provvedimento sia passato anche alla promulgazione del Presidente

effettuerò solo alcune precisazioni, perché l'intervento di chi mi ha preceduto è stato molto puntuale. Tuttavia, nella valutazione dei termini per la costituzionalità del decreto in oggetto dobbiamo svolgere alcune brevi considerazioni

urgenza del decreto-legge in quanto la mancanza di una delle sue componenti fondamentali, cioè la copertura finanziaria, comprova che sarebbe stato opportuno impiegare tempi legislativi diversi e non certo quelli del decreto.

dato il vaglio positivo al decreto-legge, ebbene penso che le motivazioni vadano cercate anche al di là di una pura e semplice contrapposizione politica: per quanto riguarda la Lega Nord e il sottoscritto infatti non possiamo che essere favorevoli ad un pronto e repentino

attraverso un decreto-legge che dimostra di per sé di non avere i requisiti di necessità ed urgenza proprio per l'assoluta incongruenza delle coperture finanziarie previste, o meglio dire non previste; se questo decreto

alle norme dell'Unione Europea tanto da giungere a questa sentenza; e addirittura questo provvedimento, nel comma 2, 2, esclude non solo i rimborsi, che vedremo quando saranno effettivi, ma l'applicabilità di questi rimborsi alle ordinarie procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto, dico che a questo decreto non solo

alle aziende che hanno fatto gli acquisti oggetto di IVA. Si crea infatti una norma ma specificatamente quelli che sono oggetto di questo rimborso non possono usufruire delle normali operazioni

con la propria scelta di voto, della astensione e di un voto contrario, l'espressione di un parere contrario essendo, come ha detto il presidente Bianco, il risultato in parità. Ma è indubbio - ed è stato riconosciuto anche dai colleghi intervenuti prima di me, anche dall'opposizione, che ricorrono tutte le ragioni di urgenza e di necessità per l'approvazione di questo decreto-legge, che consente intanto di ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee

È dunque opportuno che il Governo abbia presentato questo provvedimento e predisposto una procedura attraverso la quale dare una risposta concreta alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Si riconosce da parte di tutti l'opportunità che nel merito ci sia una trattazione e una normazione più puntuale, perché credo che a nessuno sfugga l'assoluta incongruenza della possibilità di detrarre l'IVA per l'acquisto di autovetture da turismo, ancorché intestate ad aziende che svolgono attività produttive di beni, di servizi o di altro tipo.

Quindi c'è l'esigenza di una normativa, ma a maggior ragione si deve riconoscere - e mi pare che sia stato riconosciuto - il carattere di necessità e di urgenza di questo provvedimento. Pertanto, il Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra

presidente Bianco ha richiamato quanto è accaduto ieri in 1a Commissione e

quando la Corte europea si pronuncia, perché questo di per sé spiega la necessità e l'urgenza alla base del decreto. Vedete, quando la Corte di giustizia delle Comunità europee si esprime, dichiara il diritto europeo, certifica che il principio di diritto europeo è quello che la Corte afferma, come ha fatto in questo caso. Ovviamente, nel caso di una pronuncia come quella qui considerata, la regola nazionale è incompatibile e, per la superiorità del diritto europeo che prevale, si hanno conseguenze nell'ordinamento interno. L'effetto non

di una conseguenza che tecnicamente possiamo definire come appartenente ad una fattispecie di disapplicazione: vale a dire che il giudice nazionale, chiamato a risolvere una controversia, dovrà disapplicare la regola nazionale e applicare, invece, il principio di diritto europeo, come dichiarato dalla Corte di giustizia. Quindi, dopo la pronuncia si torna nell'ordinamento interno nazionale.

incertezza del diritto. Ovviamente, in questo caso, trattandosi di una materia intrinsecamente complessa e estremamente tecnica come quella della disciplina tributaria, e, per di più, di una norma che - come è stato ricordato - stava agli atti da più di trent'anni, la situazione risultante non poteva che essere di elevata incertezza del diritto.

tutelare il cittadino contribuente, dare certezza al rapporto tra cittadino e fisco subito, togliendo subito per un profilo delicatissimo quello che era inevitabilmente un punto di elevata incertezza giuridica.

con pacatezza e serenità magari nella legge finanziaria, per fare un'ipotesi - si è preferito dare da subito la regola

non a caso, si è tradotto in un'astensione di gran parte di loro: sapendo però perfettamente che l'astensione, per il Regolamento del Senato, vale come voto contrario. Se fossimo stati alla Camera, l'espressione del voto della Commissione affari costituzionali sarebbe stata formalmente positiva, e i presupposti sarebbero stati riconosciuti. Ma qui al Senato, come è noto, l'astensione equivale ad un voto contrario e quindi i colleghi della Casa delle Libertà hanno votato per la decadenza del decreto, perché questo è l'effetto concreto al quale tendeva la loro espressione di voto. E allora, è o non è strumentale,

colleghi senatori, la Commissione affari costituzionali si è espressa dichiarando l'insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, che reca disposizioni urgenti di adeguamento ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di detraibilità dell'IVA. Non posso che esprimere il mio dissenso rispetto a quanto stabilito dalla suddetta Commissione. Ciò per una motivazione molto semplice: i presupposti di necessità ed urgenza del decreto si colgono proprio nel fatto che occorre dare immediata attuazione agli effetti della sentenza emessa in data 14 settembre 2006 e consentire, dunque, ai contribuenti di ottenere il rimborso di quanto in passato non detratto per la sussistenza di una limitazione dettata dalla normativa italiana. Tale limitazione è stata ritenuta dalla Corte di giustizia contrastante con i princìpi comunitari relativi alla detrazione. L'organismo giurisdizionale, pertanto, ne ha imposto la disapplicazione. Il decreto-legge provvede a regolare tali effetti della sentenza con urgenza, consentendo concretamente di superare le incertezze dei contribuenti in materia di detraibilità dell'IVA su determinate spese. *(Applausi

l'opposizione abbia convenuto, nei vari interventi, sulla necessità e l'urgenza di modificare questo iniquo decreto‑legge che è stato varato dal Governo.

riguarda i rimborsi dell'IVA non detratta, i quali sono stati affidati ad un canale isolato, che non comunica con i normali

giorno precedente alla scadenza della dichiarazione IVA, e quindi finisce per porre uno sbarramento ulteriore tra gli appuntamenti ordinari e la questione auto.

pochi mesi fa, la Corte di giustizia ha censurato in altra causa il comportamento dell'Italia nella restituzione della tassa società, perché erano state varate misure meno favorevoli di quelle che ordinariamente disciplinano i rimborsi. La sentenza che si riferisce alla causa, appunto la C-197/03, è stata resa l'11 maggio 2006. Nelle conclusioni censura le norme che «subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo

Proprio nel caso specifico del rimborso dell'IVA sulle auto, il Governo ha varato misure che possono essere considerate meno favorevoli rispetto a quelle ordinarie, per cui un'eventuale contestazione in ambito comunitario potrebbe esporre e certamente la esporrà - la procedura ad una nuova condanna, anche se questa potrebbe arrivare solo dopo due o tre anni dall'effettiva

di tutta la pregressa posizione IVA senza un chiarimento specifico in relazione soprattutto al tempo del rimborso dell'IVA stessa. Si potrebbero così trovare esposti ad una situazione

stabilisce che la procedura speciale non può andare avanti e comunque non può dar luogo alla compensazione. Cioè, se non ci fossero state queste zeppe poste nel decreto dal Governo, sicuramente il titolare del diritto al rimborso avrebbe potuto ad ogni scadenza

l'importo da lui dovuto dall'importo dovuto ai fini dell'IVA, e risolvere la situazione immediatamente. La nostra sensazione è che in questo modo si crei una procedura parallela rispetto a quella ordinaria, che è più favorevole al diritto ad un rimborso. Queste, signor Presidente, carissimi colleghi, sono le nostre preoccupazioni; tant'è vero che non abbiamo votato in

vista la dichiarazione di legittimità della detraibilità dell'IVA rispetto ai beni valutata in sede europea e mi auguravo che le illegittime entrate dello Stato potessero ritornare

rientrerà, come si suol dire, a babbo morto. Quindi ci troviamo di fronte alla solita fregatura e una fregatura non può essere mai urgente, né necessaria. Ne approfitto per dire che invece è urgente e necessario che venga domani in Senato il presidente Prodi, il quale oggi ha dichiarato che domani non verrà. Egli vorrà anche spiegarci

Grazie

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. Pregherei i senatori di prestare attenzione. I senatori che intendono conformarsi al parere della 1ª Commissione, e quindi riconoscere la insussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì. Al contrario, i senatori che sono favorevoli alla sussistenza di tali presupposti e requisiti dovranno votare no. I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione con procedimento elettronico.

comprendere l'orientamento della Presidenza del Senato sulla possibilità che domani si voti in merito al disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Lei comprenderà la delicatezza dell'argomento.

o se, in caso di chiusura anticipata della discussione generale, si rinvii alla settimana successiva. È una questione che pongo per poter regolare i nostri lavori.

Grazie

nuova finestra") *(LNP)*. Signor Presidente, colleghi senatori, componenti del Governo, siamo di fronte ad un provvedimento che richiede alcune riflessioni, perché è un provvedimento non di proposta, non di costruzione, non di rinnovamento o di riforma di questo Paese, ma è un provvedimento di sospensione. I cento giorni sono ampiamente passati, ci avviciniamo ai duecento e da questo Governo, da questa

di sospensione di provvedimenti già deliberati, se non addirittura proposte di abrogazione. Alcuni di carattere quasi arrogante, impositivo, come in questo caso, altri di carattere

*(LNP)*. Governare significa proporre, costruire, innovare, non significa solamente fermare, guardare indietro, rallentare o addirittura voler abrogare, voler distruggere ciò che è stato fatto in precedenza. Il metodo del cacciavite, accennato dal presidente Prodi fin dalle sue dichiarazioni programmatiche in quest'Aula, adottato poi anche da alcuni Ministri, non non porta per ora all'uso nobile di questo strumento che serve anche per costruire - soprattutto per costruire - e solo in certe situazioni

tante riforme e tanti atteggiamenti riformatori, tanti slanci che avevano dato entusiasmo a questo Paese e che erano giunti praticamente a compimento o stavano per essere

per portare questo Paese avanti verso forme di Governo più snelle, più efficienti, più europee?

da decenni si susseguono tentativi di interventi riformatori per risolvere e non più tollerare le disfunzioni che affliggono un sistema così importante come questo. Nel corso degli anni tutte le maggioranze che si sono succedute al governo di questo Paese hanno tentato di procedere a riforme settoriali, senza peraltro avere mai il coraggio di intraprendere una riforma complessiva, una riforma strategica quei cittadini che vanno messi al centro dell'azione riformatrice, dell'azione amministrativa dello Stato; quei cittadini che il ministro Castelli aveva voluto mettere in quella scritta: la giustizia si amministra nel nome dei cittadini, nel nome del popolo, come dice la nostra Costituzione; quei cittadini che devono essere al centro innanzitutto del sistema della giustizia e che chiedono efficienza, chiedono rinnovamento. Erano questi i i princìpi ispiratori di quella riforma, che posso riassumere in alcuni punti: l'ammodernamento e una maggiore attualizzazione o aggiornamento del sistema complesso della giustizia; un miglioramento del sistema di accesso alla magistratura, alla carriera di magistrato; il principio costituzionale della terzietà del giudice con la separazione delle carriere; l'introduzione di meccanismi volti a recuperare l'efficienza della professione, l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici; e, ancora, il ristabilire quel legame fondamentale tra istituzioni e cittadini, tra politica e giustizia attraverso il recupero della fiducia, della legalità, di una sana cultura e di una politica della giustizia vicina ai cittadini, superando anche quei luoghi comuni che tanto male fanno alla nostra amministrazione pubblica e alla nostra convivenza sociale e civile, che allontanano i cittadini da noi e dai sistemi amministrativi come quello della giustizia. In questo scorcio di legislatura ci apprestiamo quindi a discutere quella che può ritenersi una riforma fondamentale in questa materia, ovvero la riforma dell'ordinamento giudiziario, che non è piovuta dall'alto, che non è stata imposta, ma che ha richiesto un lavoro enorme. Ci sono voluti infatti voluti infatti oltre tre anni, quaranta mesi di discussioni, di dibattiti, di proposte, cinque letture parlamentari, un rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato, quattro astensioni dalle udienze da parte dell'Associazione nazionale magistrati e sei scioperi dell'Unione delle camere penali. Questa riforma non è quindi una riforma che è stata imposta, una riforma che è stata

ad un aggiornamento e a tener conto di quelle che sono state tutte le esigenze, tutte le componenti che hanno voluto partecipare a quella proposta.

quali norme sarebbero in vigore con questa sospensione? Le norme abrogate, quelle che, quindi, non ci sono più, o le norme che dovrebbero essere reintrodotte con una forma di riforma dell'abrogazione (non so come possa essere definita una situazione di questo genere)? Quindi quello sforzo corale dell'allora maggioranza, con la partecipazione di tutti coloro che vollero inserirsi nel dibattito e portare un contributo, ci portò ad un modello condiviso di giurisdizione, rispettoso dei princìpi costituzionali e in grado di restituire, soprattutto a quei cittadini cui accennavo prima, un servizio efficiente, un servizio in cui avere fiducia. Dopo una riflessione approfondita, nella quale in più riprese l'allora ministro Castelli è venuto sempre più incontro alle esigenze sia della magistratura, sia delle forze politiche (anche di opposizione), desta sconcerto riscontrare come ancora oggi si parli di questa come di una riforma ingiusta, che aggraverebbe l'inefficienza della giustizia italiana ed attenterebbe all'indipendenza e all'autonomia di tutti i magistrati. noi riteniamo che questa riforma rappresenti un'innovazione fondamentale in materia di giustizia, dato che, per la prima volta da oltre cinquant'anni, praticamente in tutta la nostra storia repubblicana, viene modificata la legge fondamentale in materia di ordinamento giudiziario, risalente al lontano 30 gennaio 1941. Si tratta di una riforma, quella in vigore, che incide sull'organizzazione interna della magistratura, tentando di ridisegnare il sistema di accesso in magistratura in modo tale da recuperarne la professionalità, l'efficienza, l'indipendenza e l'imparzialità. In sostanza viene a delinearsi un sistema più puntuale nella valutazione dei magistrati. A tal fine, per essere ammessi al concorso, non basta più la semplice laurea in giurisprudenza ma sono richiesti ulteriori titoli abilitanti; dovranno essere sostenuti dei colloqui di idoneità psicoattitudinale volti a valutare la predisposizione del candidato, anche in riferimento alle specifiche funzioni che egli avrà indicato al momento della domanda di ammissione al concorso; si dovrà seguire un apposito corso di formazione iniziale presso la scuola della magistratura e di seguito trascorrere i periodi dell'uditorato presso i vari uffici giudicanti, requirenti e di prima assegnazione, così che il periodo di tirocinio iniziale serva per valorizzare la formazione dell'uditore attraverso l'apporto di varie esperienze diverse. Grazie a questa riforma, finalmente anche la progressione in carriera dovrà svolgersi alla luce di profili meritocratici, venendo sganciata dal semplice avanzamento per anzianità di servizio ed affidata a momenti di effettiva valutazione (i concorsi) oltre che a corsi di aggiornamento professionale continui. In pratica, queste innovazioni cambiano la prospettiva dalla quale si deve guardare al superamento del concorso: l'essere diventati magistrati non significa più aver raggiunto un traguardo nella vita, ma un semplice punto di partenza verso una funzione che richiede costantemente impegno professionale ed aggiornamento continuo, perché il magistrato aggiornato è anche il più qualificato dal punto di vista professionale. Ma la riforma è interessante anche perché vuole garantire il principio costituzionale di terzietà del giudice, in attuazione del principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione. A tale scopo delinea il quadro della separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri, onde porre fine ad una commistione inaccettabile tra chi sostiene l'accusa e chi giudica, con la possibilità, oltretutto, di passare tranquillamente da una funzione all'altra in un modo che giudichiamo, a dir poco, inquietante. È bene precisare che la riforma proposta non sconvolge il sistema, ma prevede appunto un meccanismo che si può definire di separazione, tendenziale e di fatto, delle funzioni: pubblici ministeri e giudici continuano, entrambi, ad appartenere all'ordine giudiziario, con la differenza che, attraverso la riforma, il passaggio dalle une alle altre funzioni viene subordinato ad una serie di condizioni che si presentano come sbarramento alla continua commistione tra le stesse cui abbiamo assistito fino ad oggi. Sotto questo profilo sono stati ripetuti gli attacchi da parte del mondo della magistratura, che lamenta un vero e proprio attentato alla sua indipendenza ed autonomia. In effetti, questa critica sembra dimenticare completamente quanto sia necessario distinguere le due funzioni, in ragione della diversa professionalità che l'esercizio delle stesse presuppone. Al pubblico ministero viene infatti richiesta non tanto la cultura della giurisdizione, ma la cultura dell'investigazione, tanto spesso trascurata. della sua posizione di terzietà imposta dalla Costituzione, si richiede quella imparzialità che tuteli le garanzie fondamentali dei cittadini. Anche a livello europeo - tanto invocato in altri momenti - è sufficiente un rapido esame per rendersi conto di come la disciplina di accesso e progressione in carriera sia differente rispetto a a quella italiana. Ad esempio, in Germania si parte da un'unica formazione per tutte le professioni legali, che si articola in varie fasi e comprende esami di professionalità, al termine dei quali si sceglie una delle professioni legali. A questo punto, giudice e pubblici ministeri godono di uno *status* giuridico distinto, che continua ad essere tale per tutta la progressione in carriera. Lo stesso dicasi per la Spagna, dove la carriera in magistratura è separata da quella di pubblico ministero. Si parte tuttavia da un concorso unico per giudice e pubblico ministero, al termine del quale i vincitori scelgono tra una carriera e l'altra. Un altro risultato importante di questa riforma è la temporaneità degli incarichi direttivi (e ricordiamo a questo proposito che si tratta di un'antica rivendicazione della magistratura), oltre alla nuova strutturazione degli uffici della procura. La nuova previsione in chiave verticistica serve a recuperarne l'efficienza, individuando nel procuratore capo il compito di coordinamento della gestione delle indagini, ma anche a recuperare chiarezza, individuando il centro di responsabilità in colui che diventa l'unico titolare dell'azione penale. Con le modifiche proposte siamo sicuri che, alla fine, gli uffici di procura recupereranno l'efficienza e l'agilità gestionale che sono troppo spesso mancate al procuratore nell'organizzare i lavori degli uffici a lui sottoposti. Condivisibile è anche la chiarezza con cui viene strutturato il sistema degli illeciti disciplinari che, in tal modo, dovrebbe diventare finalmente tassativo, chiaro e indirizzato al recupero dei valori di professionalità, equilibrio, correttezza, imparzialità, indipendenza: insomma, di quella che dovrebbe rappresentare l'autonomia vera, e non meramente proclamata, per l'esercizio della funzione giudiziaria. Riteniamo che questa riforma sia stata varata, al di sopra degli interessi di parte, per rispondere ai problemi reali e contrastare l'inefficienza del sistema giustizia. E siamo convinti che, per poter fare questo, sia necessario creare un modello di magistrato più attuale e rispondente ai nuovi valori della moderna società civile, per renderlo compatibile con la richiesta di giustizia del Paese e più rispondente ai princìpi costituzionali di imparzialità ed efficienza. Un ultimo appello, anche se ora sono assenti (sono presenti solo in alcuni momenti, quelli cioè in cui è necessario il voto), lo rivolgo ai senatori a vita. Il presidente Cossiga, questa mattina, ha svolto un intervento anche condivisibile: i senatori a vita sono comunque una risorsa, per la loro esperienza e per quello che hanno rappresentato (come *ex* Presidenti della Repubblica o come personaggi della politica, del mondo imprenditoriale, scientifico, artistico e culturale).

fondamentale nella contesa tra le parti politiche; diventa antipatico per la gente, non corretto e non giusto per questa nostra Assemblea.

e che si scelga la formula della sospensione quando esistono altri strumenti normativi: le leggi si possono abrogare o si può varare una legislazione successiva, ma, comunque, non si lascia

L'intervento dell'esimio presidente Cossiga ha avuto un solo difetto: è stato svolto in un'Aula semivuota - nel momento in cui questa è stata abbandonata

bisogna essere sempre contro l'Associazione nazionale magistrati, non contro la magistratura, non contro la magistratura, perché una cosa è il sindacato e altra cosa è l'istituzione. Quel che sta avvenendo è che il Governo sta cedendo ad una forte pressione sindacale e corporativa. Ci si sta accingendo a effettuare un'operazione per cui - e mi si consentano la volgarità ed il salto - sarebbe come dire che il sistema dei trasporti non è finalizzato agli utenti, ai cittadini, ma alle esigenze dei ferrotramvieri: che le esigenze della giustizia non sono le esigenze del cittadino, ma devono partire o debbono avere il *placet* del sindacato dei magistrati, è la stessa identica cosa!

che diceva pressappoco così: «Leggi il "Corriere della Sera" e fai l'esatto contrario». L'importante è sempre avere un termine di paragone, che sia positivo o negativo, e allora, siccome quel giornale era visto come contrapposto agli interessi di un certo gruppo politico, quello era il motto che circolava a quei tempi. Oggi lo potremmo trasferire esattamente nei confronti dell'Associazione nazionale dei magistrati. Possiamo dire che sono stati risolti tutti i problemi del sistema giudiziario italiano? Possiamo dire che non esistono disfunzioni nel sistema e e nell'ordinamento giudiziario italiano? Tutti in cuor loro, e anche onestamente tanti, hanno il coraggio di affermarlo; il problema diventa il coraggio di affrontarle, perché di fronte ad un potere come quello inquirente e giudicante della magistratura, si smorzano tutte le velleità di andare a sistemare e a regolamentare un sistema che tutti, all'unisono, dicono che ha bisogno di registrazioni. È così volgare, è così sovversivo dire che per fare il magistrato bisogna superare intanto un concorso, e che non serva più la semplice laurea in legge ma magari altre prove attitudinali, che dimostrino la capacità, la predisposizione a svolgere questa delicata funzione, e pertanto stabilire che servirà anche addirittura una scuola della magistratura, così come i decreti che si vogliono sospendere hanno previsto? È così sovversivo dire che la progressione della carriera di magistrato dovrà seguire e anche o avere profili meritocratici e che non basta soltanto l'anzianità per fare carriera? Mi sembra che tutte le organizzazioni sindacali abbiano fissato termini meritocratici per distinguere all'interno di tutto il mondo lavorativo

che gli incarichi direttivi devono essere temporanei? Abbiamo troppi capi ufficio giudiziari che hanno dimostrato di non essere all'altezza del compito, ma sono ormai inamovibili! A noi sembra che la strada sia quasi obbligata. L'ultima volta che si è messo mano alla Carta costituzionale, quando si è riformato l'articolo 111 della Costituzione, mi sembra che queste Assemblee fossero interamente d'accordo nell'affermare - e lo si scrisse una infinità di volte - l'importanza della terzietà del giudice: il giusto processo in funzione del diritto ad una giusta giustizia dei cittadini! Bene, adesso dobbiamo darvi seguito. Non basta fissare princìpi; bisogna creare norme, disposizioni, dare attuazione a quanto il il Parlamento aveva ratificato. E non è forse in questa logica, in questa conseguenza il riordino degli uffici dei pubblici ministeri o la separazione delle funzioni - perché magari qui sta il nocciolo

e l'eventuale passaggio subordinato ad altre eventuali condizioni. ripetiamolo - è richiesta innanzitutto la terzietà, crediamo che al pubblico ministero sia giusto non solo chiedere che sia dotato di una certa cultura giuridica, ma anche

da tanti esuberanti procuratori, poi finiti nel nulla! Noi sappiamo come funzionano le procure e nel momento in cui vi è la fuga di notizie, qual è il ristoro che si può offrire offrire ad una vittima ormai distrutta nella propria immagine, oltre che nel proprio fisico? È così scandaloso scrivere ciò che stabilisce il

diligenza, laboriosità (termine a volte poco conosciuto), riserbo - questo forse è più deflagrante - e equilibrio e nel rispetto della dignità delle persone sottoposte alla propria alla propria funzione? Tante volte quelle stanze delle procure, che dovrebbero essere camere blindate, più che porte blindate sembravano avere porte di *saloon*, che si aprivano in tutti i sensi e più volte abbiamo letto notizie secretate e verbali

Oggi, a settembre inoltrato, a riforma partita, il Governo, sotto pressione dall'Associazione nazionale magistrati, decide di calare la scure, di bloccarla. Parliamone,

puntualizzazioni che, sotto il profilo costituzionale, rivestivano carattere di grande lezione giuridico-costituzionale per il Senato della Repubblica.

Nel momento in cui nascono conflitti tra poteri dello Stato, essendo la nostra cultura giuridica figlia della separazione dei poteri,

del privilegio di farsi portatori della sovranità popolare sono i rappresentanti liberamente eletti con mandato popolare*, ergo* i parlamentari di questa Repubblica.

Gli appartenenti all'ordine della magistratura. Possono entrare nel merito delle leggi e operare sindacato nei confronti dell'opera del Parlamento? Vi è una parte

un provvedimento e del suo contenuto: sull'*iter* e sul contenuto del provvedimento, non sul merito! Noi non possiamo accettare magistrati si rifiutino di applicare una legge perché ritenuta, nel merito, ingiusta o inopportuna;

intuire - avrebbero voluto mettere sotto un'altra parte del corpo! È possibile che la magistratura interferisca, in questo conflitto di attribuzione di poteri, con il potere che rappresenta la sovranità popolare: il Parlamento?

comportamentali: ecco perché era necessario concordare sulla responsabilità disciplinare anche degli illeciti dei magistrati, perché non esistono *legibus soluti*. I magistrati non possono essere l'unica categoria

rilasciando terroristi, che hanno reclutato altrettanti terroristi, incaricati di andare a compiere atti di violenza contro militari italiani in Paesi esteri;

Se noi sapessimo fare il nostro lavoro, non consentiremmo a questi giudici di giocare nelle pieghe dell'ordinamento giudiziario e delle leggi italiane. Visto che ho la parola vorrei lanciare un monito, che dovrà essere però seguito da un atto ufficiale, da una mozione che presenterà la Lega, sul fatto che, per evitare che terroristi vengano rilasciati, anche una volta difficoltosamente assicurati alla giustizia, da magistrati italiani, occorre trovare una formula affinché questo non avvenga più. cioè, definire ogni atto di terrorismo come atto contro l'umanità,

era l'America l'obiettivo dell'organizzazione criminale che risponde ad Al Qaeda,

penale internazionale affinché l'Italia riconosca ogni atto terroristico come crimine contro l'umanità, nessun giudice italiano potrebbe comportarsi come il tribunale di Milano.

è solo procrastinare, spinti dall'organizzazione sindacale dei magistrati. È inaccettabile. La giustizia si amministra in nome del popolo italiano.

credo che per capire bene le ragioni della sospensione non si possa prescindere dalle ragioni per cui è stato approvato questo ordinamento giudiziario. sede è stato più volte ripetuto che l'ordinamento giudiziario serve anche a rendere più celeri i processi. Ebbene, non c'è prospettiva più errata di questa. Il nostro processo penale non funziona perché il legislatore del 1988 non ha fatto una scelta precisa e decisa fra processo accusatorio e processo inquisitorio: ha preso alcune parti del processo accusatorio, le ha portate avanti, ma solamente nella parte riguardante l'indagine preliminare, il dibattimento di primo grado e non fino in fondo; poi ha lasciato assolutamente immutato il sistema delle impugnazioni, che è quello del codice del 1930. È chiaro che da una regolamentazione di questo tipo non possiamo avere che processi che durano all'infinito. A tale proposito, è bene sgomberare il campo da quello che è stato affermato da qualche senatore dell'opposizione, cioè che l'ordinamento giudiziario servirebbe anche a rendere più celeri i processi e che, quindi, la sospensione dei regolamenti di attuazione sarebbe controproducente per quanto riguarda l'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Niente di più sbagliato. L'ordinamento giudiziario è il complesso delle norme che regolano l'assunzione, la carriera, la disciplina e la preparazione dei magistrati, ma non ha niente a che fare con la celerità dei processi. Se questa fosse stata effettivamente l'intenzione del passato Governo di centro-destra, noi avremmo avuto contemporaneamente un maggiore stanziamento di fondi per la giustizia, che non c'è stato, perché per quanto io ricordi, appena il ministro Castelli ha assunto le sue funzioni la giustizia è rimasta a secco. C'erano finanziamenti per progetti finalizzati a rendere più celere la giustizia, a eliminare l'arretrato, che furono completamente aboliti. Se si prescinde dalle ragioni per cui si è arrivati all'approvazione di questo ordinamento giudiziario credo che qualsiasi argomento si porti avanti sia fuorviante. Noi abbiamo un brutto difetto, quello di dimenticare la nostra storia, il nostro passato.

come è nato questo progetto di ordinamento giudiziario, come si è portato avanti e in che modo è stato approvato. È nato perché c'era un conflitto tra la magistratura e il potere politico, esasperato da una circostanza ben precisa e cioè dal fatto che il Presidente del Consiglio del passato Governo di centro-destra era un imputato, era soggetto alla magistratura. allora, quello che si è fatto prima di arrivare all'approvazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Presidente del Consiglio (e in parte ci si è anche riusciti). Si dimentica la legge sulle rogatorie, che impediva l'utilizzazione nel processo di tutte le rogatorie, che erano il corpo principale di prova nei confronti degli imputati.

trasmissione delle rogatorie senza la necessità di autenticazione che invece quella legge voleva. Si pensò allora di fare qualcosa di più. Prima si intervenne con la legge sul falso in bilancio, che - come sappiamo tutti - è stata una sorta di depenalizzazione, di cui

giudiziario. Anche gli esponenti dell'opposizione hanno riconosciuto che il complesso di norme che rappresenta l'ordinamento giudiziario è materia di interesse comune.

con tanto vigore e con tanta chiarezza il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Mancino, senatore fino a pochi giorni fa, il quale ha

soprattutto dal fatto che il centro-sinistra ha sempre dichiarato che queste norme costituiscono un pericolo per l'indipendenza della magistratura, che è presupposto indispensabile

stranieri nello Stato italiano che sequestrano un indiziato e sorvegliato dalla polizia italiana perché sospettato di poter avere rapporti con i terroristi e che può essere una fonte di informazione

A parte il fatto che credo che il procuratore abbia questo diritto di sorveglianza, evidentemente il procuratore di Milano condivide ciò che ha fatto il suo aggiunto in materia di terrorismo. Noi sappiamo benissimo chi è Armando Spataro. Forse molti dimenticano che è quel magistrato che si è impegnato, a rischio della propria vita, ed erano pochissimi quelli che lo facevano, nella lotta al terrorismo.

che proprio i magistrati italiani hanno avuto, unici, la menzione alle Nazioni Unite per essere riusciti a battere il terrorismo senza far ricorso a leggi speciali.

per assicurare anche l'indipendenza dei giudici si commette un errore grave. Stabilire l'indipendenza del giudice quando non si assicura l'indipendenza del pubblico ministero non serve a niente, perché il giudice non avrà mai occasione di esercitare questa sua indipendenza se il pubblico ministero non gli porterà i processi in cui poter esplicare questa indipendenza.

Badate bene che quando si ristabilisce questa carriera per concorso interno, quando si dice che si agevola la carriera di chi fa i concorsi, oltre al fatto che si toglie tempo ai magistrati di occuparsi delle questioni serie per prepararsi ai concorsi, si mostra l'intenzione (perlomeno questo è il pericolo che si può generare) generare) di creare una classe di magistrati ambiziosi, che sono poi quelli più suscettibili di essere controllati quando diventano dirigenti di un ufficio giudiziario.

quanto si eliminavano gli aggiunti e si dava la facoltà di delega solo per determinati atti, accentrando tutto sul procuratore della Repubblica, facendo fare un balzo all'indietro nel tempo incredibile.

Quando, però la Cassazione, di fronte alla circostanza che non c'era alcuna ragione per spostare i processi (e, badate, non la Cassazione a sezioni semplici ma la Cassazione a sezioni unite),

che questo ordinamento giudiziario possa in qualche modo condizionare l'indipendenza della magistratura. È vero che poi si sono fatte delle modifiche, sotto la spinta e soprattutto anche per l'intervento del nostro presidente della Repubblica Ciampi, che rilevò ben quattro motivi di incostituzionalità e rimandò il provvedimento alle Camere, come è stato anche ricordato. è stato un altro segnale molto forte del fatto che si volesse comunque cercare di condizionare l'indipendenza della magistratura.

non è certamente questo il motivo. Forse uno dei motivi per cui siamo favorevoli a determinate

superiore della magistratura, che aveva istituito corsi centralizzati e corsi periferici per il miglioramento della professionalità. L'affermazione

deve uscire dalla magistratura. Come vedete, per quanto riguarda la professionalità e la capacità dei magistrati, è stata avanzata una proposta che addirittura va al di là di quello che stabilisce l'attuale ordinamento giudiziario, i cui decreti legislativi di attuazione si vogliono sospendere. Non solo. Se vogliamo poi parlare dei pericoli, diciamo allora che il vostro ordinamento giudiziario, quello che noi tendiamo a sospendere, prevede una cosa veramente incredibile: che il magistrato di prima nomina che il magistrato di prima nomina possa esercitare funzioni monocratiche, sia requirenti che giudicanti. Vi sembra veramente che possa giovare all'amministrazione della giustizia il fatto che un magistrato inesperto

se è stato trasferito è proprio perché si era dimostrato incapace di governare una procura. Se ci fosse stato l'incarico direttivo temporaneo, che la magistratura ha sempre voluto e che hanno voluto e vogliono tutti i cittadini democratici, probabilmente tutto questo non

personalmente quello che succede quando deve essere fatta una tale scelta. Ho visto la procura della Repubblica di Milano impoverirsi degli elementi migliori solo per la minaccia della separazione delle carriere; appena

Signor Presidente, indubbiamente il provvedimento di sospensione dei decreti legislativi può essere visto sotto diversi profili. vista tecnico, nel senso di un intervento che guardi alla sostanza della legge delega, a cui questi decreti legislativi attuativi danno appunto attuazione. Lo si può guardare dal punto di vista di parti in causa, che, ovviamente con competenza professionale maturata sul campo, come il collega D'Ambrosio che mi ha preceduto, svolgono delle valutazioni, anche di merito, sui concorsi, sull'opportunità, i limiti e le paure. Ho sentito dire che questa sospensione tranquillizzerà la magistratura; mi fa piacere constatare che avremo una magistratura più tranquilla, se questo deve essere un termine di paragone. lo si può vedere da un'altra angolazione, quella dei cittadini, cioè dei fruitori di questo servizio. Purtroppo, con il massimo rispetto di tutti coloro che ogni giorno lavorano nella magistratura,

più esteso del termine - ovviamente, non intendiamo solamente gli aspetti penali ma anche quelli civilistici - ci riferiamo alla formazione e alla professionalità di giudici, di pubblici ministeri e a tutte quelle norme che vadano ad incidere e ad organizzare la vita civile, sociale ed economica del nostro Paese

La pubblica amministrazione in generale può essere un elemento di supporto all'attività sociale ed economica del Paese ma può costituire anche un elemento di freno; quindi, nel momento in cui ci si confronta a livello internazionale, ci si trova con risposte, tempi e processi lunghissimi che in altri Paesi, per alcune motivazioni specifiche - per l'organizzazione ma anche per dettami costituzionali diversi - invece non esistono. Tuttavia, all'interno di questi tre aspetti, non posso non considerare che se l'esordio per una giustificazione della sospensione dell'efficacia dei decreti legislativi è quello secondo cui l'ordinamento giudiziario è stato modificato per per un conflitto esistente tra una certa parte politica e la magistratura, non posso certo credere e accettare che questa sia una risposta sufficiente per cittadini. Se la giustizia è amministrata in nome del popolo, queste non sono motivazioni condivise o condivisibili che i cittadini possano accettare.

dovuto anche al fatto che, nel tempo, mai e poi mai dal 1941 si era riusciti a portare una riforma così innovativa, pressante

incontrato in un convegno molto interessante, organizzato dall'ordine degli avvocati della Provincia vicentina, i rappresentanti degli avvocati. Un convegno a cui hanno partecipato anche esponenti locali della magistratura, dove il confronto è stato sereno e dove si sono viste le diversità di posizione. Lì è stato riconosciuto da tutti - mi sembra una ovvietà ma a quanto pare non lo è - che la situazione dell'ordinamento complessivo, ma soprattutto anche della disponibilità delle piante organiche non solo della magistratura ma anche dei servizi amministrativi, è così carente da rendere impossibile un qualsiasi efficace

ma forse per questo ho modo di vedere in maniera più disincantata quanto succede, quanti sono i problemi, quante le strette a cui è costretta la nostra comunità, i nostri concittadini quando devono rivolgersi per qualsiasi motivo alla magistratura. In quel convegno ho sentito parlare anche di organici nella mia Provincia, nella mia Regione, il Veneto, particolarmente sottodotati rispetto ad altre realtà del Paese, ma ho anche conosciuto proposte od esempi che riguardavano e si rifacevano ad altri Paesi. Paesi. Mi sono reso conto che non è solo una questione di numeri di magistrati e di personale amministrativo, perché mi sembra che la media tra numero di

(dove la sperequazione territoriale è assolutamente marcata), che è "il" problema. È un problema di normativa, un problema di approccio, un problema anche di categoria. Ulteriormente ribadisco che l'affidare ad una semplice contrapposizione con il sistema giudiziario la riforma dell'ordinamento giudiziario

tanti si riempiono bocca e su cui siamo tutti d'accordo in linea di principio, mi viene da fare una domanda: il fatto che ci siano le cosiddette toghe rosse e che la magistratura sia politicizzata, è forse una cosa che sogno io, che ho visto o letto in qualche romanzo di fantascienza politica, oppure è una realtà presente? Se diciamo che le riforme vanno fatte - e non vanno fatte contro l'indipendenza della magistratura (su questo sono assolutamente d'accordo, non si può transigere) - non si può far finta che la magistratura non abbia, essa stessa in primo luogo, violato i princìpi di indipendenza dell'istituto della magistratura. Indipendenza della magistratura non vuol certo dire

Credo che, anche se si abolisse *in* *toto* la riforma dell'ordinamento giudiziario, non verrà fatta nessuna riforma utile per

anche se si applicano ovviamente, come sappiamo, le norme in vigore nel momento in cui le questioni sottoposte a giudizio sono accadute. accadute. Il differimento di questi decreti legislativi è un'azione immotivata e direi anche pericolosa. C'era una legge approvata da questo Parlamento, una legge delega che ha generato dei decreti legislativi: differirli nel tempo - non sto tanto di differimento temporale dovuto magari ad un'esigenza oggettiva, alla preparazione o alla mancanza di alcuni strumenti attuativi - vuol dire esautorare il Parlamento di quello che ha fatto nella piena potestà della propria competenza nella scorsa legislatura. Se si voleva controriformare l'ordinamento giudiziario si doveva procedere con un disegno di legge ordinario, ma la magistratura indipendente aveva ordinato che questo non si poteva fare perché sarebbe entrato in vigore un ordinamento giudiziario nuovo, che poi magari avrebbe dimostrato di essere un buon ordinamento giudiziario: qualcuno se ne sarebbe accorto e non sarebbe stato possibile concretamente modificarlo. Vedrete che quelle lunghe pagine del programma elettorale dell'Unione sull'ordinamento giudiziario, sull'amministrazione della giustizia in generale nel nostro Paese resteranno lettera morta, soprattutto nei casi in cui andranno ad incidere sulle rendite di posizione proprie della magistratura. Quindi, chi ha violato per primo l'indipendenza della magistratura è chi ha politicizzato la magistratura, che è diventata funzionale a scelte politiche.

nel mondo della politica, però è evidente, e credo sia anche questa un'ovvietà, che la politicizzazione della magistratura abbia inciso in maniera notevole, mettendo di fronte

non ho il tempo materiale per fare una compiuta disamina del programma nella parte che riguarda la giustizia, penso di aver colto nella lettura alcune frasi generiche, di una genericità tale da far sì che ci possa stare dentro tutto o quasi tutto, sostanzialmente la volontà di abrogare l'ordinamento giudiziario riformato per tornare ad una ad una situazione anteriore e quindi, lo ripeto, ad una situazione che non è in grado di dare risposte ai cittadini nei tempi e nei modi voluti. Ho sentito parlare ancora oggi di questi aspetti, ma non ho sentito parlare di proposte concrete per migliorare il servizio ai cittadini: la parola cittadini, anzi, forse dovrebbe essere pronunciata in maniera più frequente. È scritto

Scuola della magistratura: «Dobbiamo realizzare un'efficace e rigorosa separazione di funzioni tra magistratura giudicante e magistratura inquirente, e contribuire a realizzare nel processo penale un'effettiva terzietà del giudice ed una effettiva parità tra accusa e difesa.»

uniti teoricamente nell'esprimere la necessità di dare alla magistratura una separazione delle funzioni essenziale per lo svolgimento professionale e competente nel tempo dei diversi incarichi, senza una commistione che - anche umanamente e personalmente - può essere deleteria.

sperando che non diventi una scuola succube, ma che l'indipendenza e la libertà non siano questioni di libertà d'insegnamento, di apprendimento, di crescita professionale, né siano due cose distinte o contrapposte. Ma ecco quello che mi preoccupa in questa frase (e riprendo a leggere quanto è scritto nel programma dell'Unione): «in modo da rafforzare una cultura unitaria, cui devono ispirarsi la magistratura inquirente, quella giudicante e l'avvocatura».

cui, in maniera molto rigida, la magistratura inquirente, quella giudicante e l'avvocatura devono avere una certa forma mentale, determinata dagli indirizzi impressi nella

l'ordinamento giudiziario, probabilmente anche la riforma che è stata varata non sarà in grado di per se stessa di fornire quella scossa - anche se la potrà avviare - necessaria alla nostra alla nostra strutturazione giudiziaria, affinché il debito pubblico giudiziario si contenga e si riduca. Partire, però, dal presupposto che il mondo della giustizia, a trecentosessanta gradi, debba avere una cultura unitaria, credo sia da stigmatizzare in quanto elemento portante che ci fa comprendere le motivazioni vere e profonde per cui vengono proposte la sospensione dei decreti legislativi e quindi l'attuazione compiuta della riforma dell'ordinamento giudiziario. *(Applausi*

Signor Presidente, onorevoli senatori, potremmo dire che quest'Aula rappresenta una situazione

intervenire in assenza dell'interessato. Sono

dal tono ammaliante e quasi suadente supportati da un linguaggio e da una capacità tecnici pari al livello professionale del senatore. Il senatore D'Ambrosio ha voluto dirci

Mastella, che trae origine da necessità tecniche.

implicite» nella cosiddetta legge Castelli, approvata dal Parlamento il 25 luglio 2005.

Con una certa disinvoltura, con l'atteggiamento di chi ha sempre la chiave della verità, tipico del

dal fatto che all'epoca dell'elaborazione del provvedimento Castelli, che è durata qualche anno nella scorsa legislatura, vi era il Presidente del Consiglio dei ministri sotto giudizio.

fra il Presidente del Consiglio, che giocava a fare il topo, e un gruppo di magistrati - non la magistratura - che giocavano a fare il gatto.

esperienza professionale nella città di Milano, conosco le qualità del dottor D'Ambrosio, ne conosco anche la rettitudine e la serietà, però questo non lo salva, non lo esime dal "vizietto" che comunque anche il magistrato composto, integerrimo, preparato e intelligente può concedersi, perché è uno *status* quasi di superiorità intellettuale, forse anche umana, a certi livelli. Egli può concedersi la libertà di dire che le motivazioni tecniche che sottendono il provvedimento di iniziativa del sono volte a modificare e frenare gli inconvenienti tecnici recepiti dalla legge Castelli, la quale sarebbe riconducibile ad una sorta di barricata nei confronti della posizione dell'ex Presidente del Consiglio. E per rendere credibile la cosa, con maestria e con capacità tecnica che non può essere la mia nel campo giudiziale,

solo in funzione di quel topo particolare che doveva salvarsi dal gatto, come dicevamo prima. Ha ricordato la legge sulla rogatoria ed altro; ha richiamato finanche, e con ciò suscitando una mia sorpresa - perché ne conosco il tratto di discrezione e di ristrettezza dell'uomo

il famoso dottor Spataro, rappresenta il punto più alto dell'indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero e che qui la riforma Castelli del luglio 2005, andando a toccare le disposizioni che regolamentano la figura e l'ufficio del pubblico ministero, avrebbe commesso

di ledere l'indipendenza del pubblico ministero. Signori, amici intimi, senatori, signor Presidente, in realtà qui ci stiamo interessando delle seguenti materie perché la legge Castelli non altro tratta che dell'accesso alla magistratura, della progressione economica e della funzione dei magistrati, delle competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici, della Scuola superiore della magistratura, del tirocinio e formazione degli uditori, dell'aggiornamento professionale, del Consiglio direttivo della cassazione e altro ancora, tutto di natura strettamente ed unicamente ordinamentale. Allora il volere, come è normale fare nelle persone abili, ampliare il confine dell'argomento di cui si discute così da realizzare una grande confusione e far emergere un dato assolutamente inveritiero, anzi falso, perfido ed ingannevole, secondo cui da una parte ci stanno sempre e soltanto i buoni e dall'altra ci sono soltanto i cattivi;

a subire questa sorta di trattamento, per cui non ci scandalizziamo e non ci meravigliamo.

a cos'è chiamato il Parlamento, a cosa sono precostituiti i due rami del Parlamento se non - come diceva qualcuno di cui abbiamo reminiscenze storiche e culturali - a svolgere attività in favore del prossimo e della collettività? Che cos'è, amici, la politica, la gestione della politica e la politica nelle istituzioni,

Diciamolo chiaramente: il programma dell'Ulivo comprendeva l'indicazione che la legge Castelli sarebbe stata tolta di mezzo.

Ma non si può prendere l'istituzione per i fondelli. Qui si pretende di prenderci per i fondelli. Non si può, attraverso una cosiddetta sospensione dell'efficacia, disporre l'abrogazione di fatto della legge. Si passi dalle Si passi dalle Aule, si decida l'abrogazione della legge! Noi sappiamo, signor Presidente, che con molto meno le leggi cadono in desuetudine; già la sola a lungo scarsa o saltuaria applicazione

subentra alla legge scritta la cosiddetta legge materiale, cioè l'uso costante di una norma che viene applicata in sostituzione di quella scritta. Pertanto,

che è indicato nel programma elettorale dell'Ulivo attraverso la via surrettizia della sospensione, ovvero del congelamento *sine die*. Infatti, non è vero che si congelerebbe per un anno, perché questo è il primo passaggio. Penso che un Governo che adotta questa più che scarsa sensibilità, questa ostilità, questo senso di arroganza nei confronti dell'opposizione, ma direi anche nei confronti di se stesso, quantomeno di larga parte dei suoi componenti, sia un Governo